Tra l'altro, proprio per evitare strumentalizzazioni, era stata vietata la riproduzione per stralci delle interviste. Nell'ambito di tali interviste, nella parte non pubblicata, il direttore rilevava che l'istituto del servizio civile nazionale si configura quale modalità di difesa della Patria con mezzi ed attività non militari: quindi, difesa della Patria non armata. Sempre nell'ambito di tali interviste, il direttore dell'Ufficio sottolineava che il servizio civile fornisce ai giovani «un'opportunità di donare un anno della propria vita alla Patria, al servizio del prossimo e a loro stessi poiché diventa un'occasione unica di formazione e di crescita personale». In particolare, il direttore affermava che il destinatario principale dei progetti di Servizio civile è proprio il giovane Noi avevamo fatto lo slogan: «Il servizio civile cambia la tua vita e cambia la vita degli altri», che è stato stampato anche su un francobollo celebrativo del servizio civile nazionale, proprio per enfatizzare questo momento di formazione civica del giovane volontario, che prima costruisce il suo rapporto con la collettività, con le istituzioni e i principi costituzionali e poi lo mette al servizio degli altri. Quindi, da tali dichiarazioni, emerge come dottor Borea, abbia voluto rappresentare l'esperienza del servizio civile come forma di adempimento volontario del dovere costituzionale di difesa della Patria, intesa quale esperienza volta a favorire la crescita di una consapevolezza civica nei giovani e a formare un cittadino migliore, attivo, consapevole dei suoi diritti e cosciente dei suoi doveri verso la collettività; un cittadino che sappia relazionarsi con le istituzioni in modo corretto e nel pieno rispetto delle regole democratiche. Pertanto, appare chiaro che l'esperienza del servizio civile non è uno strumento di politica sociale (lo vedremo più avanti), come peraltro qualcuno vorrebbe farlo diventare. Peraltro, anche nella parte dell'intervista in cui è stato affermato che il servizio civile sopperisce ad alcune carenze del settore pubblico di assistenza ai meno fortunati, è palese l'intenzione di riferirsi a quelle situazioni in cui il cittadino non percepisce la piena presenza dello Stato, e perciò l'intervento del servizio civile è finalizzato, in un'ottica ampia di difesa non armata della Patria e anche di coesione sociale interna, a rinsaldare i legami tra i cittadini e le istituzioni, là dove la fiducia nei confronti di queste ultime sia venuta meno. In particolare, occorre segnalare che le situazioni in cui tale fenomeno è maggiormente sentito sono quelle dove si verificano forti disagi, sia collettivi che individuali, per esempio nelle categorie dei disabili e dei grandi invalidi (la sospensione della leva obbligatoria, ad esempio, ha fatto venir meno la possibilità per i ciechi di guerra di avere accompagnatori, servizio oggi in parte supplito dai giovani volontari del servizio civile nazionale), oppure quando ci sono state situazioni di grande gravità (subito dopo il terremoto all'Aquila, i giovani del Servizio civile nazionale che hanno aderito all'invito sono affluiti in città per i primi soccorsi).

il servizio civile interviene per contribuire alla tenuta delle istituzioni, anche attraverso la presenza dei suoi volontari quali punti di riferimento in situazioni di criticità e disagio estremo. Ciò avviene anche all'estero: anche recentemente, scrivendo al Capo dello Stato, ho fatto presente che i giovani del servizio civile sono in Kosovo, Albania, Israele, Giordania e Libano; sono in 60 Paesi del mondo, dove curano, insieme ai giovani militari (con funzioni naturalmente diversificate), aspetti che riguardano le missioni di pace all'estero, in questo caso non con le armi ma con funzioni di rapporto con la popolazione civile.

crediamo, del servizio civile nazionale. Ricordo - e ne approfitto per fare un appello, perché siamo al Senato - che da quasi due anni il Governo ha presentato un disegno di legge di riforma del servizio civile. Tale servizio è nato nel 2001 con 180 volontari il primo anno,

E poiché la legge prevede che il Fondo nazionale sia alimentato dallo Stato, ma anche dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle fondazioni (oggi, purtroppo, sostanzialmente è lo Stato a contribuire), quando anche le Regioni contribuiranno (alcune lo fanno già),

Sembra anche importante che venga dopo la seduta di martedì pomeriggio, quando il Governo, con il sottosegretario Davico, ha accettato di considerare che, per le prossime scadenze referendarie, anche il personale delle ONG possa votare dove già votano i militari impegnati nelle missioni internazionali di pace. Registro quindi una somma di aperture molto positive.

nonviolento dell'obiezione di coscienza, cioè di coloro che rifiutano l'utilizzo delle armi. È importante che siano seduti ad uno stesso tavolo, perché

nelle date indicate dall'interrogante (25 febbraio e 31 marzo), il Comitato si è riunito il 14 giugno, il 1° luglio, il 12 novembre e il 14 dicembre: Si segnala inoltre che il 28 dicembre 2010 si è riunito il gruppo di lavoro sulla sperimentazione, composto da alcuni membri del suddetto Comitato, incaricato di svolgere specifica attività di studio connessa alla realizzazione di un progetto per la sperimentazione della difesa civile non armata e nonviolenta. Con riferimento invece alla somma stanziata a favore delle attività di ricerca e sperimentazione di nuove forme di difesa civile non armata e nonviolenta svolte dal Comitato, si segnala che nel documento di programmazione finanziaria elaborato dall'Ufficio nazionale per il servizio civile per l'anno 2010 è stato previsto un finanziamento (a valere sul Fondo nazionale per il servizio civile) di 100.000 Tuttavia, si fa presente che tale somma non si è potuta impiegare, in quanto nel corso del 2010 il Comitato ha svolto prevalentemente funzioni propositive di nuove iniziative, sempre rientranti nell'ambito di competenza, piuttosto che attività di ricerca. Al riguardo, occorre segnalare che le attività svolte dal Comitato sono state rivolte alla programmazione di varie iniziative, che sono state poste all'attenzione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile al fine di valutarne la validità e l'interesse. Considerato, tuttavia, che non è stato possibile realizzare nel 2010 alcuna di tali iniziative, le risorse stanziate in tale anno sono state riconfermate per l'anno 2011, sia per l'attuazione delle iniziative stesse sia per l'attività di ricerca.

su come potrebbe essere una convivenza tra Forze armate e Difesa civile nazionale nel momento in cui si trattasse di organizzare queste forme di difesa civile non armata e nonviolenta. È una delle questioni che potremmo inserire anche nella riforma, al fine di valorizzare al massimo il lavoro di questo Comitato che, ripeto, è già importante di per sé: che siano seduti allo stesso tavolo ufficiali delle Forze armate

presentati all'Ufficio nazionale per il servizio civile. Con il primo quesito si chiede di conoscere se l'Ufficio nazionale per il servizio civile abbia o meno intenzione, in vista della valutazione dei progetti per il 2011, di modificare la prassi finora seguita circa le modalità di comunicazione agli enti sulle limitazioni imposte in sede di valutazione, prevedendo che le stesse vengano rese note contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di merito provvisoria dei progetti, anziché successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva. Secondo l'interrogante tale diversa modalità di comunicazione consentirebbe agli enti di presentare eventuali osservazioni prima della conclusione del procedimento, così come previsto per i rilievi riguardanti i punteggi attribuiti ai progetti. Al riguardo si precisa che il procedimento di valutazione dei progetti è disciplinato dal «Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi», stessi», approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2009, che, al paragrafo 4.4, prevede un subprocedimento volto all'acquisizione da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile delle osservazioni, formulate dagli enti, in ordine ai punteggi attribuiti ai progetti. Gli enti in tale fase possono visionare i punteggi attribuiti ai progetti, anche in relazione alle singole voci della scheda progetto, e confrontarsi, in piena trasparenza, con l'amministrazione su particolari aspetti della valutazione. Tale subprocedimento ha lo scopo di ampliare il principio di partecipazione degli interessati al procedimento, nell'ambito di una procedura definita concorsuale dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3956 del 2006. La ragione che ha indotto l'amministrazione a non estendere tale subprocedimento ad ulteriori eventuali osservazioni, diverse da quelle relative ai punteggi risponde all'esigenza di non appesantire la procedura di valutazione dei progetti stessi, allungandone eccessivamente i tempi di conclusione. Peraltro, occorre segnalare che la prassi di comunicare agli enti, con apposito provvedimento, le limitazioni da apportare ai progetti successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, non viene a ledere il diritto degli interessati alla partecipazione al procedimento di valutazione, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa. Infatti gli enti possono presentare la richiesta di accesso agli atti del procedimento, con le modalità previste dalla legge n. 241 del 1990. Sulla base di tali considerazioni, l'Ufficio nazionale per il servizio civile non riscontra, allo stato, motivi validi per modificare l'attuale procedura. Riguardo al secondo quesito, con il quale si chiede di conoscere il numero degli enti che hanno presentato osservazioni in merito ai punteggi ai progetti compresi nella graduatoria provvisoria, si segnala che all'Ufficio nazionale per il servizio civile sono pervenute osservazioni riconducibile a 40 enti, relative a 513 progetti, corrispondenti a circa il 20 per cento di quelli presentati. Con riferimento al terzo quesito, con il quale l'interrogante intende conoscere quante delle osservazioni presentate dagli enti siano state accolte, si forniscono i seguenti dati: 1.660 sono le osservazioni pervenute all'Ufficio nazionale per il servizio civile; 236 sono quelle accolte, pari a 129 sono i progetti per i quali è stato modificato il punteggio precedentemente attribuito. Si segnala infine che in molti casi è stata presentata più di un'osservazione sullo stesso progetto. si segnala inoltre che il numero dei progetti finanziati con il bando del 3 settembre 2010 per i quali è stato modificato il punteggio a seguito delle osservazioni pervenute è pari a 19, per complessivi 187 volontari. Riguardo all'ultimo quesito, con il quale l'interrogante chiede di conoscere se l'Ufficio nazionale per il servizio civile intenda modificare la prassi volta ad acquisire le osservazioni presentate dagli enti in ordine ai punteggi, poiché tale misura avrebbe un limitato impatto sui punteggi attribuiti in origine, si osserva quanto segue. Come si è già rappresentato, il procedimento di valutazione dei progetti è disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2009, che prevede una fase in cui è possibile da parte degli enti formulare osservazioni in ordine ai punteggi attribuiti ai progetti. Ciò consente all'Ufficio nazionale per il servizio civile di rilevare eventuali errori di valutazione, con l'obiettivo di sanare gli stessi ed evitare disparità di trattamento. Quanto alle perplessità espresse dall'interrogante circa il limitato impatto di una siffatta misura, si fa presente che le osservazioni inoltrate dagli enti hanno riguardato soltanto il 20 per cento dei progetti valutati nel 2010. Appare quindi evidente che, a fronte di una bassa percentuale di enti interessati a presentare eccezioni, l'incidenza delle modifiche apportate ai punteggi non poteva che risultare esigua, tenuto conto peraltro che molte delle osservazioni pervenute erano prive di fondamento. Si ritiene che ben più preoccupante sarebbe stata la situazione se le eccezioni e le osservazioni presentate dagli enti fossero state fondate ed avessero portato ad uno sconvolgimento della graduatoria, in quanto un'ampia revisione dei punteggi sarebbe un sintomo evidente di un'attività di valutazione dei progetti superficiale e disattenta. L'esiguità delle osservazioni rappresenta, al contrario, un indicatore indiretto della correttezza e linearità delle valutazioni effettuate dalla Commissione. Un altro indicatore della correttezza dell'operato della Commissione, nonché dell'efficacia della procedura, si evince dalla drastica riduzione del contenzioso.

Peraltro, per due di tali ricorsi, il TAR del Lazio, nella fase cautelare, si è pronunciato favorevolmente all'amministrazione. Pertanto, si è orientati a confermare la procedura finora seguita anche in occasione della valutazione dei progetti per il 2011, in quanto rispondente ai principi di buona amministrazione e trasparenza. che esiste un problema di fondo, perché se la coperta continua a restringersi, è evidente che il rapporto tra i progetti presentati e quelli accolti diventa sempre più esiguo, anche se i progetti hanno un punteggio tale per cui negli anni passati sarebbero stati ammessi al finanziamento. Quindi, c'è la frustrazione e l'avvilimento di enti, anche dei giovani, che vorrebbero partecipare al servizio, ma che si vedono impediti a farlo. a farlo. Noi consideriamo un valore i quasi 300.000 giovani che hanno fatto il servizio civile nazionale: costoro non solo hanno svolto un anno di attività, ma vanno a costituire un'amplissima riserva di volontariato. Tantissimi di loro hanno espresso in tutti i sondaggi e le rilevazioni indipendenti un grande tasso di soddisfazione per il lavoro svolto, diversamente dall'obiezione di coscienza, dove inevitabilmente, a causa degli enormi numeri, i ragazzi venivano mandati a svolgere attività anche avvilenti, non gratificanti

andando ad ingrossare il numero di coloro che in Italia svolgono questa attività fondamentale. Ad esempio, quelli che sono addestrati a fare servizio civile

economica di risorse sufficiente ogni anno per far corrispondere la volontà dei giovani di partecipare a questo servizio, la progettazione sempre più raffinata degli enti e la possibilità di dare soddisfazione e di far fare quest'esperienza a tutti coloro che in effetti vogliono dedicare un anno della loro vita al servizio degli altri.

La cosa importante è che tutto il processo sia molto trasparente e che quando, a seguito

l'interpellanza parlamentare di cui discutiamo è stata firmata da 34 senatori - quindi un numero abbastanza consistente -sia dell'opposizione, sia della maggioranza. Osservo, intanto, che l'interpellanza giunge alla discussione e alla risposta dopo un anno e mezzo dalla sua presentazione; in altre materie, in altri contesti, su altri problemi, probabilmente questo lungo periodo avrebbe comportato l'automatico decadimento

sappiamo si riferisce alla situazione di una regione a noi molto vicina, il Kosovo, dove l'evoluzione dei contrasti e dei conflitti tra le varie etnie e i rapporti conflittuali hanno uno sviluppo estremamente più lento di quanto non avvenga nelle altre aree di crisi. Il problema è quello della salvaguardia della minoranza serba in quella regione, a causa anche della mancata integrazione nel Paese. Un'integrazione che naturalmente non c'è, anche perché la stessa non ha alcuna intenzione di procedere lungo questa strada. di questi contrasti sono note a tutti: sono ragioni che trovano le radici in secoli di odi e di conflitti, e la situazione è molto delicata, anche se i disordini verificatisi nel marzo del 2009, dopo la dichiarazione d'indipendenza del Paese, naturalmente sono una pallida immagine di quelli accaduti in passato. Il problema, andando nel concreto, è quello della salvaguardia della minoranza serba, soprattutto nel settore che storicamente è sempre stato sotto il controllo del nostro personale militare (mi riferisco all'area occidentale del Kosovo, quindi alla minoranza serba nella regione concentrata nell'abitato di Gorazdevac), e della salvaguardia dei luoghi di culto che in quella regione sono particolarmente importanti: il patriarcato di Pec e il monastero di Decani. Io ho avuto il piacere di incontrare qui a Roma

che ha salvato finora quei luoghi di culto, stava (parlo del 2009) progressivamente diminuendo; diminuzione che, naturalmente,

per la salvaguardia di questi luoghi, non ritenga che si debba comunque fare qualcosa, pur nell'ambito

devo dire all'interpellante che francamente anch'io, che ho ricevuto le carte, sono rimasto perplesso nel dover rispondere ad un'interpellanza del 26 novembre 2009.

il rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite in Kosovo, che guida la missione UNMIK dell'ONU, per quanto ridotta nelle sue dimensioni, è ancora il nostro ambasciatore Zannier.

Ne cito almeno due. Il primo riguarda le elezioni amministrative che si sono tenute l'anno scorso nella zona Sud del Kosovo (lasciamo stare la parte Nord, Mitrovica, che ovviamente, come l'interpellante sa, mantiene ancora una netta separazione, non solo etnica, ma anche amministrativa e politica rispetto alla cosiddetta parte Kosovo). Ebbene, nella zona Sud, là dove ci sono delle minoranze serbe, queste hanno partecipato al voto amministrativo, e addirittura abbiamo - credo di non sbagliare - tre Comuni c'è stata un'apertura.

nell'area kosovara, ma, anch'esso è avvenuto senza incidenti, sia per il senso di responsabilità del patriarcato, che non ha fatto manifestazioni, al di là di quelle normalmente consentite, sia per la grande attenzione prestata dalle stesse forze

2, sostanzialmente c'è stato il ritiro delle truppe dal territorio e il loro insediamento, le basi, sono oggi di pronto intervento, rispetto a quella che era la presenza precedente. Senza fissare date, in

del nostro contingente è strettamente legata, in termini numerici, alla questione della presenza complessiva di KFOR.

voleva la presenza di un'organizzazione multilaterale che ufficialmente e formalmente si occupasse della questione.

di cambiamento della situazione in Kosovo sia avvenuto. Purtroppo, le difficoltà stanno poi nel sistema parlamentare e di governo. Come sapete, è stata contestata l'elezione del Presidente e c'è stata una difficoltà ad individuarne c'è un sistema parlamentare ancora molto frantumato, molto diviso e c'è questa strana caratteristica per cui la minoranza serba, che in base alla Costituzione ha diritto ad avere alcuni seggi nel Parlamento di Pristina, si trova al momento al Governo, cioè fa parte della maggioranza.

la forte attenzione del Governo italiano e della comunità internazionale, così come la preoccupazione che questo processo di dialogo tra Serbia e Kosovo sia

dei soldati italiani che nel 1943 facevano lo stesso lavoro che stanno facendo i soldati italiani in questo momento, a dimostrazione del fatto che, purtroppo, l'odio

alcune questioni. Innanzitutto, la situazione nel Paese continua a suscitare forte preoccupazione, perché non si registrano fatti innovativi. Voglio ricordare, ad esempio, che moltissimi esponenti della cosiddetta Onda verde sono ancora in carcere, vi sono state pesanti condanne e che le condizioni detentive di questi detenuti sono assolutamente fuori da ogni *standard* accettabile a livello internazionale. Ricordo, altresì, che gli stessi *leader* dell'opposizione, Moussavi e Karroubi, sono agli arresti domiciliari

e di attivisti dei diritti umani. La maggior parte dei *media* non allineati al regime sono stati chiusi, così come gli uffici dei principali partiti politici riformisti. Quindi, la situazione non ha segnato alcuno spazio virtuoso per poter fare una valutazione diversa da quelle fatte in precedenza.

al traffico di stupefacenti, stranamente a seguito di accuse iniziali di insurrezione contro lo Stato. Quindi, anche questo credo faccia riflettere sulla situazione in Iran. Come Governo italiano, ovviamente, in seno all'Unione europea ed alle Nazioni Unite abbiamo sempre sostenuto ogni misura, ogni presa di posizione volta a promuovere il rispetto delle libertà fondamentali in Iran e quindi dei diritti umani. Tra le più recenti iniziative, ricordiamo la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 12 aprile 2011 con cui sono state adottate misure restrittive (divieto di ingresso e congelamento di eventuali beni posseduti nei Paesi membri dell'Unione europea) nei confronti di 32 esponenti del regime ritenuti responsabili di gravi violazioni dei diritti civili. Abbiamo anche sostenuto l'approvazione, da parte della Terza Commissione dell'Assemblea Generale dell'ONU,

gli astenuti. Vorrei anche ricordare che gli iraniani - ironia della sorte - hanno accolto 23 raccomandazioni che nel corso dell'esame periodico universale sulla situazione dei diritti umani tenutosi a Ginevra, presso il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, facciamo all'Iran. Due di esse sono state formulate su iniziativa dell'Italia per sollecitare la ratifica della Convenzione contro la tortura e sul bando delle esecuzioni di minori in accordo con l'articolo 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Sottolineo ancora il fatto

il Consiglio diritti umani per il mandato 2010-2013 e la mancata elezione di un rappresentante di Teheran nella Commissione ONU sulla condizione femminile. Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha anche approvato la nomina di un relatore speciale incaricato di verificare la situazione dei A questo punto dobbiamo dire che il Governo condivide l'opinione prevalente in sede dei Paesi membri dell'Unione europea secondo cui denunce e misure sanzionatorie non possono essere fini a se stesse, ma servono ad indurre le autorità iraniane a impegnarsi per migliorare le condizioni dei diritti umani e ad aprirsi al dialogo con la comunità internazionale. È ovvio che vi deve essere anche una forte azione di pressione politica. Peraltro, noi crediamo anche che ancora avviare una serie di misure parallele, soprattutto con contatti diplomatici regolari, con corsi di formazione e seminari di taglio accademico, con esperti dentro e fuori dell'Iran, per mantenere vivi dei canali di comunicazione con una realtà che viene preclusa alla comunicazione ed ai rapporti normali internazionali, per avere anche opportunità di rappresentare le nostre preoccupazioni per i casi di violazione più urgenti ed eclatanti, nel tentativo almeno di salvare alcune vite umane. In questo senso, l'approccio dell'Italia nella difesa dei principi resta fermo e allo stesso tempo aperto al dialogo per svolgere pressione e persuasione allo stesso tempo. Peraltro, devo dire che la situazione in Iran è in via di evoluzione, almeno così sembra, sul piano politico, per le notizie che possiamo cogliere.

poi una presenza anche di altri attori. Altrimenti, questo apparato minaccia di diventare autoritario e dittatoriale anche in senso di monopolio economico ancor di più contribuendo a non creare alternative e possibilità di dialogo con la società civile iraniana. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Mantica per aver interpretato in senso ampio l'interrogazione, presentata parecchio tempo fa e ispirata ad un episodio preciso riguardante il regista Panahi.

Ritengo estremamente importante che l'azione che il Sottosegretario ci ha illustrato continui e che non ci si lasci scoraggiare dai risultati

poiché è chiaro che fintanto che le pressioni sono unicamente esterne non è verosimile un qualche progresso significativo. Sottolineo, cogliendo l'occasione della replica a questa interrogazione, un caso ulteriore. Il sottosegretario Mantica ha citato l'attività, per mantenere

sotto l'egida della Commissione per la condizione delle donne delle Nazioni Unite. Credo sia particolarmente importante un'azione specifica del Governo al riguardo, perché non è davvero tollerabile che la partecipazione a un'attività, che per l'appunto va nella direzione che lei, Sottosegretario, ci ha indicato, di mantenere contatti e di portare avanti operazioni non direttamente politiche, ma di carattere culturale,

usata come accusa nei confronti di una cittadina di quel Paese. Credo sia opportuno poi manifestare solidarietà a tutti coloro che sono in carcere e subiscono violenze e restrizioni della libertà personale per essersi battuti per i diritti umani, per la democrazia e per la libertà in quel Paese. È estremamente importante che il Governo cerchi con ogni mezzo di far sentire una forma di solidarietà, anche se certamente è molto difficile, a tutti coloro che sono impegnati in questo senso.

(ECOSOC), uno degli enti destinati a raccogliere i problemi relativi all'uguaglianza di genere, al miglioramento della condizione della donna nel mondo, alla promozione dei diritti delle donne in campo politico, economico, civile e sociale: in questo organo da un anno figura l'Iran. La domanda è sempre la stessa: come possono avvenire fatti del genere? Avvengono non per scelta politica, ma per meccanismi procedurali che portano a situazioni irritanti come questo, ma che comunque regolano la vita delle Nazioni Unite. Infatti, nel caso specifico delle elezioni per i membri della Commissione sulla condizione femminile, che hanno avuto luogo il 28 aprile del 2010 (infatti, l'interrogazione della senatrice Carloni è del maggio, quindi poco dopo i fatti), sono stati rinnovati 8 seggi per il mandato 2011-2015. Al gruppo Asia, cui appartiene l'Iran, erano riservati due seggi, per i quali si sono candidati due Stati, l'Iran e la Thailandia. A fronte di tale circostanza, dal momento che si trattava di un'elezione non competitiva (due candidati per due

e, da ultimo, nel periodo 2006-2010. Quindi, ha semplicemente continuato ad esserne membro. Dunque, l'elezione del 2010 di cui parliamo era il prolungamento di un periodo quadriennale che aveva visto l'Iran già membro della suddetta Commissione. Queste sono purtroppo le norme e le prassi che regolano il funzionamento di tale organo delle Nazioni Unite, ma di casi abbastanza irritanti di questo tipo ne abbiamo trovati anche in altre strutture. Voglio ricordare la Commissione diritti umani, che poi si è trasformata per cercare di evitare

che prevedono appunto che nel caso in cui il numero dei candidati sia limitato, non essendoci una votazione e quindi una selezione, si vada in automatico. Va comunque ribadito con forza, lo abbiamo detto prima e lo ripetiamo, che la tutela e la promozione dei diritti delle donne in Iran, come in tutti gli altri Paesi dove la dignità femminile sia calpestata, rappresenta una delle priorità della politica estera italiana dei diritti umani, o dei diritti della persona, come giustamente precisava il Presidente questa mattina in occasione di un altro dibattito, e che il Governo italiano è costantemente impegnato su queste materie anche in seno, peraltro, a questa Commissione sulla condizione femminile di cui abbiamo parlato. L'Italia ha sostenuto attivamente la risoluzione di condanna per la situazione dei diritti umani in Iran, approvata peraltro il 21 dicembre dall'Assemblea generale dell'ONU, e, da ultimo, quella approvata dal Consiglio dei diritti umani a Ginevra, che, come ho detto prima in risposta al senatore Malan, ha nominato un relatore speciale dell'ONU incaricato di elaborare un rapporto sulla situazione dei diritti umani in Iran.

Tuttavia, vorrei osservare il fatto, spiacevole per così dire, che questa interrogazione, presentata all'indomani

molto colpita. Sembra veramente grottesco che la Repubblica islamica dell'Iran, fondata proprio sull'oltraggio, l'offesa e la discriminazione delle libertà delle donne (la Repubblica dei *mullah* è questo) e che ogni giorno si macchia di reati gravissimi, da questo punto di vista

che sembra essere stata arrestata l'11 maggio, quindi qualche giorno fa, a Shiraz, nella provincia di Fars in Iran. Secondo fonti riferite all'Aidos (associazione

si fa carico per manifestare pesanti critiche, è sostanzialmente inattivo, cioè è stato bloccato. Si tratta di un

mira ad acquisire il controllo dei centri di protezione delle donne che sostituirebbero in questo caso le ONG che fino ad ora, tra l'altro, hanno anche realizzato tali centri. Credo che a tutti sia chiaro cosa ciò voglia dire in un Paese come l'Afghanistan in cui la condizione della donna,

lo *shock* e la tragedia, magari verrebbe condannata o indicata al pubblico ludibrio. Anche per l'acceso dibattito sviluppatosi nella comunità internazionale, cui ha partecipato pure il Governo italiano, il progetto è fermo e finora non ha prodotto effetti. Il testo è stato, infatti, sottoposto al gruppo di lavoro per la riforma della legge penale in cui siedono esperti dei maggiori donatori. Pur riconoscendo l'utilità di talune proposte, di talune proposte, quali l'istruzione elementare obbligatoria per le donne e l'utilizzo della polizia femminile per gli interrogatori, il gruppo ha ampiamente emendato il testo. Quali sono i punti più critici di questa proposta di regolamento? Il potere del Ministero degli affari femminili di nominare i direttori dei centri (anche quelli gestiti da ONG); la notifica alla polizia di ogni donna ammessa nei centri; la possibilità di escludere la donna dal centro se accolta da parenti, indipendentemente dalla sua volontà; la mancanza di norme sulla *privacy*; il divieto di uscire dal centro per le donne ivi rifugiate; l'obbligatorietà di esami medici; la canalizzazione dei fondi a favore delle case rifugio nel bilancio del Ministero degli affari femminili. La versione rivista dai donatori e dalle agenzie internazionali attribuisce al Ministero degli affari femminili solo un ruolo di supervisione, mantiene l'indipendenza gestionale e finanziaria dei centri gestiti da ONG e lascia la scelta e l'applicazione dei criteri di ammissione alla direzione dei centri. ONU, ambasciate, *media* e ONG hanno condotto un'intensa campagna di sensibilizzazione per spingere il Governo afghano ad accettare le modifiche proposte. Il progetto di regolamento, peraltro, è ancora all'ufficio legislativo del Ministero della giustizia afghano. Da parte nostra, continuiamo a seguire con attenzione questo problema. Colgo l'occasione - anche se siamo molto pochi in Aula, ma di occasioni non ne abbiamo molte - per dare qualche idea di quello che è l'impegno italiano in materia in Afghanistan. dal 2001 ad oggi il sostegno a progetti a favore delle donne afghane da parte dell'Italia ammonta a 15 milioni di euro. Circa la metà dei fondi stanziati sono andati ad Herat e vedono la popolazione femminile come beneficiaria diretta

abbiamo promosso la costituzione presso la procura generale di Kabul di un'Unità per la repressione dei reati contro le donne, consentendo l'emersione di vicende che sarebbero rimaste impunite; partecipiamo ad un progetto per favorire le pari opportunità da parte delle istituzioni afghane; sosteniamo il Centro di risorse per le donne in politica; finanziamo l'attuazione del Piano d'azione per le donne del Governo afghano, l'iniziativa di UNIFEM per la protezione delle donne più vulnerabili, il progetto di UNFPA per la promozione della salute riproduttiva, il programma di formazione e sviluppo dell'imprenditoria femminile; lo scorso 8 marzo ad Herat è stata inaugurata una nuova struttura per le donne costruita dalla cooperazione italiana. Voglio anche ricordare che il 24 e 25 maggio si terrà a Roma una conferenza sull'attività di una rete di ONG, la cosiddetta Afghana, che sta operando anch'essa in maniera autonoma, solo con un contributo parziale del Governo italiano, in questa materia. A seguito della promulgazione da parte del presidente Karzai della famosa legge che sul diritto di famiglia, per coloro che aderivano o sono aderenti allo sciismo, discriminava nei confronti delle donne, ricordo che l'Italia ha immediatamente agito attraverso i propri canali di dialogo con il Governo e per il tramite degli organismi multilaterali, fornendo anche una completa analisi del testo legislativo ed esprimendo preoccupazione per le norme legislative *in itinere*. L'intervento italiano, in raccordo con quello internazionale, ha consentito peraltro un'ampia revisione della legge, una regolamentazione che in ogni caso rappresenta un passo avanti rispetto all'assenza di norme che consentiva di richiamarsi alla cultura molto restrittiva della Il processo di ricostruzione dell'Afghanistan procede a passi molto lenti. È un cammino irto di ostacoli che richiederà, soprattutto nei settori dei diritti della donna e dell'amministrazione della giustizia, molto tempo, impegno e grandi risorse. In gioco ci sono complesse dinamiche, tribali e religiose e consolidate pratiche tradizionali. In Afghanistan persistono fenomeni dolorosi: stupri, delitti d'onore, matrimoni forzati. Ma si registrano - e dobbiamo dirlo con forza - anche segnali positivi:

però mi permetta di esprimerlo pubblicamente): lei sarebbe un ottimo Vice Ministro alla cooperazione internazionale se facesse parte di un Governo che avesse a cuore questi temi, avesse fatto una riforma della legge sulla cooperazione allo sviluppo e avesse deciso di impegnarsi con una spesa maggiore di quella attualmente prevista per le missioni. Signor Sottosegretario, sono uno dei 15 colleghi che non partecipano al voto sulle missioni, però come vede, continuiamo a interessarci, e non lo facciamo a fasi alterne, in quanto apprezziamo lo sforzo che viene fatto. Lo apprezzeremmo ancora di più se nella copertura

da noi paventate siano bloccate e che il nostro Governo sia fermo nel mantenere una posizione sulla democrazia che tenga conto della libertà delle donne in ogni parte del mondo, della libertà dei generi in ogni parte del mondo e quindi della possibilità di scegliere le regole che si danno.

anche se alcuni di noi ritengono che forse dovrebbe essere il motivo predominante, e spereremmo (ma questo tutti: non abbiamo il privilegio della coscienza) che questo possa essere il modo in cui esportiamo la democrazia, diciamo, mondo. Concludendo, la ringrazio delle informazioni. Sono in massima parte soddisfatto, e le auguro di riformare anche il settore della cooperazione allo sviluppo, con tutto quello che ne consegue.